La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1º agosto. Resta confermato che nella giornata di oggi saranno discusse le mozioni su sicurezza del trasporto ferroviario, G8 e promozione energia solare. Per quanto riguarda le mozioni sul G8, saranno oggetto di discussione le mozioni Dini, D’Alia, Bricolo, Pinotti, Marinaro, Pedica e Peterlini. I tempi delle tre discussioni generali saranno armonizzati al fine di consentirne la conclusione entro la seduta antimeridiana. Le dichiarazioni di voto e il voto avranno luogo nella seduta pomeridiana di oggi, che inizieraalle ore 17 anziche´ alle ore 16. Seguira poi l’esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunitaparlamentari. La relazione della Giunta sul caso Castelli, come gia stabilito, saradiscussa nella seduta antimeridiana di domani. Si ricorda che le iscrizioni a parlare in discussione generale dovranno pervenire entro le ore 19 di questa sera. La votazione, per la quale e richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, avraluogo con le modalita giacomunicate, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 8-bis, del Regolamento (votazione nominale elettronica nella seduta antimeridiana e successivamente possibilita di comunicare il proprio voto ai senatori Segretari fino alle ore 19). Nella giornata di domani fino alla seduta antimeridiana di giovedı23 luglio saranno esaminati il rendiconto e l’assestamento del bilancio dello Stato, nonche´ i documenti definiti dalla Giunta eventualmente non conclusi oggi pomeriggio. Per quanto riguarda la seduta pomeridiana di domani, le votazioni non avranno inizio prima delle ore 17,30. Le interrogazioni a risposta immediata, gia previste per la seduta pomeridiana di giovedı23 luglio, avranno luogo – a causa della indisponibilita del Governo – in altra data. La seduta sarapertanto dedicata agli altri La prossima settimana, la discussione generale e le repliche sul Documento di programmazione economico-finanziaria si svolgeranno nella seduta pomeridiana di lunedı 27 e nella seduta antimeridiana di martedı28 luglio; le dichiarazioni di voto e la votazione della risoluzione nella seduta pomeridiana dello stesso giorno. Per la discussione di rendiconto e assestamento e del DPEF, rispetto alla consueta ripartizione proporzionale, i tempi saranno ripartiti tra i Gruppi tenendo conto delle esigenze rappresentate dai Gruppi di opposizione, attraverso cessioni da parte dei Gruppi della maggioranza. Nel prosieguo della settimana prossima si passera poi alla discussione del decreto-legge recante misure anticrisi, attualmente all’esame della Camera dei deputati. Il calendario al momento prevede sedute, se necessario, fino alla mattina di sabato 1º agosto. La concreta organizzazione della discussione del provvedimento e` peraltro rinviata alla prossima Conferenza dei Capigruppo, non appena saranno definiti i tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.